di Ilva. Ieri Franco Bernabè, audito alla Camera dei deputati nella Commissione attività produttive, ha detto con grande chiarezza che non ci sono più i soldi per pagare le forniture del gas. Io credo che sia arrivato il momento della verità e della chiarezza in merito al tema di Ilva. Ricordo che in ballo ci sono 20.000 posti di lavoro. La vicenda Ilva è giunta alla sua crisi più grave e quindi merita attenzione da parte di quest'Aula e anche una comprensione piena dell'indirizzo che il Governo vuole assumere sulla vicenda. Ci sono dati che parlano per noi: la produzione è ai minimi storici, migliaia di lavoratori in cassa integrazione, impianti in degrado, assenza di investimenti... *(Brusìo)*. Scusate, colleghi, capisco che 20.000 posti di lavoro possano non essere al centro della vostra attenzione, ma al centro della nostra ci sono e quindi siete pregati di avere un minimo di serietà in questa vicenda. questa vicenda. Abbiamo la necessità di capire perché il processo di decarbonizzazione è bloccato, a che punto si trova la vicenda del piano industriale di questa importante realtà produttiva, alla quale peraltro è collegato tutto il sistema produttivo italiano e non solo italiano. Noi abbiamo atteso; avevamo detto in quest'Aula, già in tempi non sospetti, che gli interventi del Governo sarebbero stati finalizzati a

in condizioni gravi. Ecco, quel tempo è arrivato con le parole dure come pietre di Franco Bernabè. Chiedo, allora, che prima di ogni altra questione, Presidente, lei riferisca al Governo la volontà di quest'Aula di discutere in merito al piano industriale, di discutere dell'atteggiamento di ArcelorMittal rispetto agli investimenti in questa azienda e del futuro di lavoratori, tanti lavoratori, che aspettano una risposta dalle Istituzioni, a Genova come a Taranto, sapendo che in ballo non c'è solo il già importantissimo futuro di Ilva, ma quello della serietà e della struttura industriale del nostro Paese.

che lo stabilimento in passato aveva una potenzialità di produzione fino a 8 milioni di tonnellate; quest'anno scenderà a 3 milioni di tonnellate. Come è noto, c'è la presenza dello Stato e la presenza di un azionista privato, ma tutti i progetti che darebbero prospettive sia all'impianto sia al territorio (penso al tema della decarbonizzazione, dell'elettrificazione della produzione, della produzione di reduced iron*), sono avvolti nella più totale incertezza. Nel frattempo c'è una situazione di emergenza che riguarda le forniture di gas, che a fine ottobre si interromperanno. L'azienda, stando alle dichiarazioni del presidente Bernabè, audito ieri presso la Commissione attività produttive della Camera, non ha le risorse per garantire la continuità produttiva - perché di questo stiamo parlando - di un impianto che dà lavoro a migliaia di occupati, da cui dipende il resto del gruppo e una parte molto importante del sistema manifatturiero italiano. A questo punto, stante la gravità della situazione che mette a rischio migliaia di posti di lavoro diretti e dell'indotto, le prospettive di quell'impianto, di quelli di Genova, di un intero territorio che dipende in misura significativa dalle prospettive industriali dell'ex Ilva, chiediamo che il Governo si assuma fino in fondo le proprie responsabilità.

cosa ha intenzione di fare il Governo per le prospettive industriali della ex Ilva di Taranto e degli altri stabilimenti del gruppo in Italia; cosa ha intenzione di fare il Governo, inoltre, per garantire la compatibilità ambientale della produzione siderurgica nell'area di Taranto, la continuità dei progetti di decarbonizzazione, che richiedono ingenti risorse pubbliche, la continuità di una grande realtà produttiva del Paese che non può essere abbandonata al proprio destino.

fatto di poca rilevanza; è fondamentale, invece, che le persone possano andare a lavorare, da una parte in sicurezza e dall'altra anche con la speranza che la loro attività produttiva abbia un futuro e una continuità.

e dell'associazione «Octavia», che assistono ai nostri lavori.

che tali sentenze si riferiscono anche al superamento dei valori limite in Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Quindi non si evince la motivazione di restringerla solo a quattro Regioni.

questione che riguarda molte città, in particolare la capitale d'Italia. Vorrei cogliere l'occasione di questa dichiarazione di voto in merito all'emendamento in esame per formulare

la circolazione dei veicoli nella città di Roma. Chi parla ha fatto azioni molto forti per cercare di implementare il trasporto pubblico nella nostra Capitale:

metro C, infrastruttura che deve collegare il Sud e il Nord della capitale d'Italia, perché crediamo fermamente che al cittadino si debba dare la possibilità di scegliere il trasporto trasporto pubblico. Se è vero però che esiste un diritto alla salubrità dell'aria costituzionalmente sancito, lo è altresì che esiste un altro diritto costituzionalmente sancito, quello alla libera circolazione delle persone e noi non possiamo bloccare la circolazione a circa 800.000 romani. Questo provvedimento entrerà in vigore il 1° novembre, quindi ci corre l'obbligo veramente di appellarci al sindaco Gualtieri per fargli comprendere che ci vogliono logica e attenzione nella valutazione di interventi di questo genere.

Colleghi, diamo per acquisito che il chiacchiericcio che supera di poco anche il bisbiglio rende impossibile seguire i lavori anche alla Presidenza, da qualsiasi lato dell'Aula provenga. Quindi, per cortesia, cerchiamo di moderarci.

dell'idea di portare avanti tutte le politiche per incentivare il trasporto pubblico locale. Abbiamo presentato un emendamento per aggiungere risorse al trasporto pubblico locale e ne abbiamo presentato un altro per aggiungere risorse al *bonus* trasporti. Stiamo cercando di convincere

prima della data del 1° ottobre 2025. Siamo ad ottobre 2023. Il Governo sta impedendo alle Regioni di essere virtuose in via autonoma e di provvedere a favore della tutela della salute dei residenti prima della data stabilita dal Governo stesso. Forse non è chiaro che noi stiamo parlando non solo della limitazione alla circolazione dei veicoli intesa come una seccatura per gli utenti della strada: noi stiamo parlando di una misura che è dettata da un problema gravissimo, relativo alla tutela della salute delle persone. Non so se sapete che in Italia muoiono 60.000 persone a causa dell'inquinamento atmosferico molte di più si ammalano, soprattutto nelle Regioni del Nord coinvolte da queste sentenze. Nella sola Lombardia muoiono ogni anno 15.000 persone a causa dell'inquinamento; nella città di Milano ne muoiono 1.500. Ora, a fronte di un problema di questo genere, che riguarda la tutela e la sopravvivenza delle persone, fissare un termine prima del quale non è possibile per le Regioni legiferare nel senso della riduzione mi sembra veramente un affronto agli italiani che vivono in quelle zone e rischiano ogni giorno la vita.

al problema dell'inquinamento, prima di prevedere dei divieti - come giustamente anche voi sottolineate - bisogna incentivare il trasporto pubblico locale. Ma bisogna mettere risorse per il trasporto pubblico locale. Noi chiediamo che ci siano risorse per il trasporto pubblico locale e vi chiediamo di votare a favore del trasporto pubblico locale.

azione venga intrapresa nella direzione dell'abbassamento dei limiti di inquinamento dell'aria non può non prendere in considerazione e sottolineare che debba essere fatto senza ulteriore consumo di suolo, senza impermeabilizzazione dello stesso, nel rispetto degli *habitat* naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica. Si rischia altrimenti che, per mettere una toppa, si crea un buco ben più grosso, con danni all'ambiente e alla qualità dell'aria.

valutata l'inammissibilità di molti emendamenti dell'opposizione che non ha fatto storie e non li ha ripresentati per l'Aula, perché esulavano dal contesto delle quattro Regioni di cui si interessa il decreto-legge in oggetto. In questo caso parliamo di un emendamento che va a che va a individuare soluzioni specifiche per le funivie di Savona, con il commissario già nominato, e via dicendo. Vorrei semplicemente segnalare quest'anomalia, perché evidentemente è sfuggita alla Presidenza.

condivisa o meno, sul fatto che non è esattamente lo stesso emendamento, per cui è stata fatta una valutazione in questo senso. Peraltro, c'era comunque un parere contrario anche della 5a Commissione su tale emendamento. Questa è la valutazione che aveva fatto la Presidenza. In ogni caso, la ringrazio per la segnalazione.

all'articolo 1-*ter*. In pratica si parla dell'aeroporto di Malpensa, sempre in Lombardia, sempre in quella zona

il trasporto merci su gomma sia altamente inquinante - ed è assolutamente vero - e che, per ridurre l'inquinamento, sia una buona cosa trasferire il trasporto merci per via aerea. aerea. Sappiamo tutti che gli aerei elettrici ancora non li abbiamo visti in giro, o almeno non sono comunemente utilizzati. Pertanto, il trasporto aereo in realtà continua a insistere sull'innalzamento delle soglie di inquinamento. Quindi sarebbe sicuramente meglio trasferire il trasporto merci, piuttosto, su ferro. Ma che cosa accade a Malpensa? C'è stata una decisione del Ministro dell'ambiente e della Commissione di valutazione di impatto ambientale che ha decretato che l'allargamento del sedime aeroportuale, che teoricamente doveva andare a occupare la brughiera che contorna l'aeroporto di Malpensa, non è una scelta condivisibile né ammissibile e, quindi, l'aeroporto di Malpensa non si può allargare. Questo secondo il Ministro dell'ambiente

modifica al testo in pratica si vuole riconoscere il carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell'intervento sull'ampliamento del traffico merci. Attenzione, quindi, perché questo è un trabocchetto. Io tifo per il Ministro dell'ambiente su questa decisione,

al processo che ha portato a presentare il piano futuro per uno scalo come Malpensa, che deve evidentemente conciliare l'aspetto legato allo sviluppo sostenibile, quello dell'occupazione e anche quello dell'impatto ambientale

del rispetto dell'ambiente, puntando quindi a un modello di sviluppo sostenibile. Dichiarare sito di interesse strategico Malpensa oggettivamente è una scelta importante, perché prende atto che quella è la porta principale anche del cargo italiano verso l'esterno, in una zona, quella lombarda, nel Nord del Paese, che è una di quelle che esportano di più a livello europeo. Mettere in condizioni Malpensa di poterlo fare, è sicuramente positivo. Quello che chiediamo è che ciò venga fatto, però, nel rispetto dell'intesa già raggiunta fra Regione Lombardia e i Comuni del sedime, che hanno compiuto un lavoro molto prezioso. Se fosse approvata la modifica proposta dalla maggioranza, senza tenere conto del lavoro fatto dalla Regione Lombardia, guidata dal centrodestra, e dai Comuni del territorio, che prevede una serie di compensazioni ambientali e azzera questo tipo di lavoro, dando mandato pieno alla società aeroportuale di riprendere il progetto originario, si rischia veramente di svilire e mettere a repentaglio un lavoro prezioso fatto da amministratori di centrodestra e di centrosinistra e dalla Regione Lombardia. Invito quindi il centrodestra a ripensarci, perché probabilmente non sa di questo lavoro: basterebbe alzare il telefono e chiedere al presidente Fontana. Perdono comunque un'occasione e rischiano di non valorizzare al meglio il lavoro che è stato fatto dai territori. Sono sempre molto attento a quello che fanno i territori, che tengono conto dell'esigenza di conciliare - come dicevo prima - il diritto all'occupazione, il mantenimento degli investimenti, ma anche il rispetto dell'ambiente.

Quindi, va bene continuare a presentarlo, ma vorremmo capire anche perché il Governo non risponde favorevolmente alle richieste di questo ordine del giorno. solo per specificare il fatto che continuando a votare ordini del giorno siamo convinti che il Governo presto inserirà le richieste

Signor Presidente, colleghe e colleghi, l'inquinamento atmosferico è un subdolo nemico della nostra salute. È invisibile, insidioso, agisce in modo lento e silenzioso e i suoi effetti a lungo termine sono implacabili. In Italia d'inquinamento atmosferico si muore: questo è un dato tangibile. Il nostro Paese in Europa detiene il triste primato per il numero di decessi prematuri annui.

Il nostro Paese in Europa detiene il triste primato per il numero di decessi prematuri annui causati da polveri sottili e da particolato aerodisperso. Il dato è sconvolgente: parliamo di 60.000 decessi annui, ossia circa 140 morti premature al giorno. è ignorare il problema, rassegnarsi alla sua esistenza e accettarlo come un inevitabile danno collaterale del nostro vivere moderno. Grave e dannoso è insistere nel non intraprendere, anche intenzionalmente, concrete azioni di contrasto che possano utilmente mitigare gli effetti dell'inquinamento e favorire un'aria più pulita e sana.

Come dicevo, l'inazione climatica è un fatto grave e irresponsabile per cui ognuno di noi, forse inconsapevolmente, sta già pagando un caro prezzo in termini di salute e qualità della vita. Questa situazione si sta aggravando tanto che la qualità dell'aria in tutta Italia continua ulteriormente a peggiorare. Da diverse settimane le stazioni di monitoraggio dell'ARPA in diverse Regioni italiane stanno segnalando un costante superamento dei livelli di particolato sottile, raggiungendo in alcuni casi livelli fino a dieci volte superiori a quelli raccomandati Il 12 maggio 2022, l'inazione del Governo ha portato la Corte di giustizia europea a condannare l'Italia per aver superato in maniera sistematica e continuata il valore limite annuale fissato per il biossido d'azoto

Il 13 settembre 2023 è stato approvato dall'Europarlamento il testo di revisione della direttiva europea sulla qualità dell'aria, che fissa norme più stringenti per allineare gli *standard* europei con le linee guida dell'OMS e raggiungere un ambiente privo di inquinamento nocivo entro il 2050. Noi oggi ci limitiamo a discutere solo e unicamente della semplice conversione in legge di un decreto-legge utilizzato nuovamente come stratagemma per tamponare il rischio di incorrere in un'altra infrazione comunitaria. Il provvedimento in discussione è infatti completamente insufficiente per il rientro nei limiti emissivi necessari a garantire agli italiani il diritto alla salute, e non risponde neppure appieno alle richieste della Corte di giustizia europea. Non c'è traccia infatti di una concreta pianificazione o programmazione strategica di medio-lungo periodo per decarbonizzare tutti quei settori responsabili dell'inquinamento atmosferico. Insieme a molte associazioni e organizzazioni che hanno espresso le loro perplessità su questo atto del Governo, ci associamo all'appello di incrementare con urgenza gli sforzi per una seria e credibile politica di riduzione dei principali fattori inquinanti. Bisogna intervenire immediatamente sui settori dei trasporti, dell'energia e dell'industria, responsabili di oltre il 60 per cento delle emissioni di ossido di azoto. Particolare attenzione va posta sull'ammoniaca prodotta dall'industria agrozootecnica, un inquinante che finora è stato poco considerato nelle normative, ma che costituisce il fattore principale della formazione di particolato sottile. Abbiamo bisogno di piani per la qualità dell'aria non solo aggiornati, ma soprattutto incisivi e monitorati, che possano orientare i finanziamenti verso attività economiche a basso impatto ambientale. Pensiamo solo alle maggiori risorse economiche da impegnare per il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, settore da elettrificare in modo completo e veloce; oppure al potenziamento delle politiche a sostegno della mobilità attiva, in particolare per gli spostamenti su scala urbana e per l'intermodalità della ciclabilità con tutte le categorie di trasporto collettivo, ma anche alla progressiva eliminazione dei sussidi per l'acquisto di automobili endotermiche o ibride, a vantaggio dei soli veicoli elettrici. Vanno liberate risorse economiche per incentivi ambientalmente favorevoli da destinare all'acquisto di biciclette di ogni categoria in regola con il codice della strada. Vi è anche la necessità di promuovere una pianificazione strutturata e sistemica, che preveda misure organiche per la riduzione della domanda di mobilità. Tali misure devono agevolare l'utilizzo del vettore ferroviario rispetto alla scelta dell'intermodalità ferro-gomma e accelerare l'ammodernamento delle flotte delle imprese di autotrasporto. Abbiamo bisogno di maggior coraggio, di maggiore responsabilità e soprattutto di un forte spirito innovativo da parte di questo Governo, che invece, anche per l'adeguamento agli *standard* comunitari sulla qualità dell'aria, si limita a ricorrere all'istituto del decreto-legge, che non garantisce in modo tangibile la possibilità di godere di un'aria sana e respirabile, bene comune per tutte le persone. Ribadiamo che la programmazione strategica deve prevedere: il potenziamento di infrastrutture di trasporto che consentano una comoda e più economica mobilità ai cittadini, disincentivando di contro l'utilizzo costoso dell'auto privata; il potenziamento di opzioni di trasporto che consentano lo spostamento su ferro e non su gomma; interventi risolutivi in agricoltura e in allevamento per limitare le emissioni di ammoniaca. Il mondo fuori da quest'Aula, la società, le nuove generazioni e l'economia chiedono al Governo e alla politica di agire subito e di adottare urgentemente politiche concrete di riduzione delle emissioni. La ciliegina sulla torta di questo provvedimento di mero adeguamento alla sentenza di condanna della Corte di giustizia europea è data infine dallo stravagante subemendamento presentato all'ultimo minuto, che prevede - e lo cito testualmente - di riqualificare aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e di valorizzare il turismo all'aria aperta. Non esiste alcun nesso logico che giustifichi un subendamento di questo genere con il tema della qualità dell'aria, né nella realtà dei fatti, né nella risposta ambigua ed evasiva dei suoi proponenti. Ecco, se sono queste le vostre misure più efficaci per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, allora vuol dire che nel Governo tira davvero una brutta aria. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo serietà e coerenza. Chiediamo di uscire dal *tunnel* di miope paralisi e di insopportabile inazione in cui ci ha ricacciati questo Governo. Chiediamo di trasformare i propositi di mitigazione e di adattamento climatico in azioni vere e reali. Per questo motivo, annuncio il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

in premessa, per richiamare nuovamente l'attenzione di questo Governo sul suo ricorso smodato - e, francamente, immotivato - alla decretazione d'urgenza. Evidentemente non sono bastate le parole del presidente Mattarella, che ha invitato il Governo a cessare di fare ricorso a questo tipo di strumento; soprattutto, ha invitato, nel momento in cui si fa ricorso alla decretazione d'urgenza, almeno a mantenere una omogeneità dei provvedimenti, a non inserire norme eterogenee, a non affastellare nei testi normativi norme che si riferiscono ad ambiti diversi. Questo lo ribadisce anche l'operatore del diritto, l'avvocato, che poi, quando si trova a dover applicare queste leggi, deve fare i conti con un testo eterogeneo, inservibile per certi versi o, comunque, molto spesso contraddittorio, perché non è sistemico nella creazione della norma. Ciò impone la necessità, prima ancora di parlare del provvedimento odierno, di riflettere anche sulla funzione e sulla natura di questa Camera. Il Senato insieme alla Camera dei deputati compongono il Parlamento, che è un organo legiferante: significa che le leggi deve farle, non ratificarle. Noi,

senza poter discutere; spesso non possono essere presentati emendamenti o, se vengono presentati, c'è un termine così stringente da non poter essere neanche esaminati.

è capitato anche in altre occasioni) alla correzione in Assemblea di espressioni semantiche, di allocuzioni, di terminologie, di definizioni, come se non ci fossero gli uffici preposti a questo scopo, come se non ci fosse nessuno che si occupa effettivamente di scrivere leggi e noi ci presentassimo in questa mi dispiace dirlo - approssimativa. Questo non è possibile, non lo possiamo assolutamente accettare. Fatta questa premessa, dolorosa ma necessaria, sulla quale mi auguro che il Governo voglia fare finalmente una seria riflessione, passando all'esame del testo, non posso che esprimere ovviamente la distanza del nostro Gruppo da questo modo di da questo modo di approcciare il problema ambientale. Ma davvero vogliamo credere che stabilendo una proroga di un anno alle disposizioni europee sulla limitazione delle emissioni si aiuterà l'ambiente, si risolverà il problema ambientale? Questa mi ricorda molto, signora Presidente, la proroga al termine di scadenza delle concessioni balneari. Mi sembra più o meno la stessa situazione: siccome non sappiamo come gestirla, e ci sono degli interessi precostituiti e diffusi, buttiamo la palla oltre la linea d'angolo e poi vediamo quello che accade. Non funziona così. Non basta una proroga di un anno per dire che il problema ambientale si risolverà. Non basta semplicemente un approccio defaticante per dimostrare che il Governo veramente si vuole impegnare per l'ambiente. Soprattutto non basta e non lo possiamo accettare, quando in questo stesso anno abbiamo assistito a a fenomeni climatici estremi e a veri e propri stravolgimenti del nostro territorio, che richiedono non soltanto provvedimenti precisi, ma anche una maggiore attenzione e una programmazione di lungo termine per affrontare il problema dell'emergenza climatica. Per tutti questi motivi, ovviamente, il nostro voto non può che essere contrario, perché non è questo il modo in cui si approccia l'ambiente, non è questa la tutela che chiediamo al Governo di avere nei confronti della tematica ambientale. Per questo motivo, a nome del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope, annuncio il voto contrario.

conversione di un decreto-legge che porta la firma del nostro ministro Pichetto Fratin, per mettere al passo l'Italia con le disposizioni in materia di inquinamento, con particolare attenzione alla qualità dell'aria. Il rischio era quello di incorrere in sanzioni pecuniarie, previste dalle infrazioni aperte nei confronti del nostro Paese dalla Corte di giustizia europea. Rischio che ora viene scongiurato attraverso l'adeguamento delle norme e della loro ricaduta sulle prescrizioni che sono di competenza dei territori. In particolare, gli allarmi riguardano le Regioni più produttive della nostra Nazione: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna devono ora aggiornare i propri piani di qualità dell'aria. È evidente come sulla qualità dell'aria pesi il fatto che queste Regioni sono il motore produttivo del nostro Paese. Le fabbriche tendono a inquinare sempre meno, ma purtroppo emettono ancora fumi inquinanti. Attorno alle fabbriche e ai distretti produttivi ruota un traffico veicolare di merci e servizi del terziario, che contribuisce ovviamente a peggiorare il livello qualitativo dell'aria. le prescrizioni del presente decreto riguardano anche la circolazione stradale e i mezzi che possono circolare. Il traffico, in particolare dei mezzi a gasolio, è quello che viene posto sotto osservazione e limitato, in quanto emana i più alti valori di PM10 e di ossido di azoto. Le limitazioni dovranno riguardare il traffico urbano, ma anche quello extraurbano, posta la grande concentrazione di auto anche sulle arterie principali. Il passaggio a veicoli sempre più prestanti dal punto di vista ambientale (gli euro 5 e gli euro 6) riduce le emissioni inquinanti medie e ci porta a veicoli a maggiore sostenibilità ambientale. L'altro obiettivo che ci poniamo e che dobbiamo perseguire è quello di incentivare il trasporto pubblico e la facilità di utilizzo, da parte dei cittadini, di mezzi pubblici efficienti. Il percorso è quello che è stato delineato dal "Fit for 55": una graduale sostituzione dei mezzi in circolazione più inquinanti con mezzi più affidabili dal punto di vista ambientale. Il Governo intende adottare una serie di misure per avvicinarsi all'obiettivo europeo e quindi prosegue il monitoraggio dello stato dell'ambiente, il controllo delle fonti di inquinamento e l'adozione di misure per ridurre l'emissione dei principali inquinanti. Siamo consapevoli che non è solo un obiettivo *green*, ma anche un obiettivo di salvaguardia della salute dei cittadini italiani. L'Italia deve quindi fare la sua parte e la sta facendo, posto che il quadro è comunque in deciso miglioramento rispetto ai picchi negativi di inquinamento atmosferico. La maggioranza di centrodestra ha a cuore la qualità dell'ambiente. Fatevene una ragione, amici della sinistra: non è un vostro monopolio. Attraverso un lavoro di squadra con le Regioni e l'attento lavoro del Parlamento la maggioranza ha presentato modifiche puntuali al decreto-legge, mettendo a punto dispositivi per superare le criticità ambientali evidenziate in sede europea. Questa è una tappa di un percorso iniziato da tempo. Ad esempio il mio Piemonte, in questi ultimi tre anni, ha dimostrato, con rilevazione certificata dall'Agenzia regionale per l'ambiente, l'efficacia delle misure messe in campo, finanziate con fondi regionali e nazionali. Ha triplicato le risorse per il miglioramento dell'aria, ha dato sostegno alle famiglie per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, ha stanziato aiuti per le aziende al fine di sostituire i mezzi più inquinanti, ha rottamato 704 autobus inquinanti e 749 seguiranno nel 2024, ha stanziato 9 milioni di incentivi regionali per sostituire stufe e impianti di riscaldamento inquinanti. Su questo decreto purtroppo in Commissione una collega ci ha dipinti come assassini. Voglio ricordare che il PIL europeo rappresenta circa il 25 per cento di quello mondiale; cioè un quarto della ricchezza mondiale è prodotta in Europa. Dall'altra parte, per produrre questa ricchezza l'Europa immette nell'atmosfera il 6,4 per cento dei *greenhouse gas* mondiali. Questo dato fa capire che l'Italia e l'Europa sono già virtuose rispetto al resto del mondo. Certo, si può fare di più, dobbiamo farlo e lo faremo, ma sapendo rispettare le peculiarità di ogni Stato europeo. È quello che chiediamo anche per lo stop ai motori termici e per le case *green*: una gradualità che, salvaguardando l'obiettivo dell'abbattimento dei *greenhouse gas*, salvaguardi anche la nostra economia, le nostre imprese, il lavoro dei cittadini e la ricchezza delle famiglie italiane. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole di Forza Italia. *(Applausi)*.

fatto riferimento a dei dati, ma sinceramente non so quale sia la sua fonte. A me, viceversa, risulta che nell'ultima settimana nella città di Milano sono stati superati i valori delle emissioni nocive di ben 10 volte i limiti consentiti dall'Organizzazione mondiale della sanità; altro che miglioramento, la situazione è in precipizio.

si perdono uno-due anni di tempo nei quali le Regioni virtuose potrebbero intervenire meglio e prima di quanto il Governo stia imponendo loro. si sta respirando una pessima aria. Il provvedimento al nostro esame se la sta prendendo comoda di fronte ai gravi rischi per la salute collettiva derivanti dall'esposizione agli inquinanti atmosferici, la cui pericolosità è riconosciuta ormai da decenni da parte di studi sempre più numerosi e accreditati. Si dimentica che nonostante qualche miglioramento riscontrato in Europa a seguito dell'introduzione delle normative e le misure di contrasto europee, respiriamo ogni giorno in un Paese tra i più inquinati d'Europa. Vi è un'area - quella della Pianura padana, da cui la sottoscritta proviene, vivendo a Milano in particolare - che registra l'aria peggiore dell'intera Unione europea. Un terzo di chi vive in queste Regioni respira aria inquinata da particelle invisibili quanto pericolose presenti in misura estremamente superiore ai limiti fissati. La circolazione delle autovetture concorre chiaramente al superamento di queste soglie. Secondo l'elaborazione di Openpolis dei dati Eurostat in Italia muoiono più di 60.000 persone l'anno; 15.000 persone muoiono in Lombardia, 4.000 nella città metropolitana di Milano, 1.500 nella città di Milano. A questi dati dobbiamo aggiungere coloro che si ammalano di gravi patologie, quali il cancro e malattie gravissime alle vie respiratorie.

lo posticipa. Quindi noi avremo ancora un anno di tempo affinché le Regioni provvedano a limitare la circolazione e un altro anno affinché questi limiti vengano inseriti nel piano d'aria. In questi due anni però quelle 15.000 persone in Lombardia continueranno a morire. È per questo che mi è stato detto che io vi ho tacciati di essere degli assassini, anche se chiaramente non ho usato questo termine: ma 15.000 persone in Lombardia che muoiono ogni anno dovrebbero dovrebbero rappresentare un'urgenza e quindi il Governo anziché porre un limite prima del quale le Regioni non possono legiferare, dovrebbe fissare una scadenza entro la quale hanno l'obbligo di farlo, ma se sono virtuose, possono farlo prima. del provvedimento, non ci si riesce a rifornire del materiale che serve per le batterie delle macchine elettriche. Ma stiamo scherzando! Tutta l'Europava in questa direzione e ce la fa, solo l'Italia evidentemente non ci riesce. Il problema, però, è che deve essere sostituito il trasporto pubblico; deve essere utilizzato il trasporto pubblico per gli spostamenti delle persone, quindi bisogna aiutare i Comuni ad andare in questa direzione. Le Regioni devono aiutare i Comuni. Milano non non è male a livello di trasporto pubblico. Certo, mancano i parcheggi di interscambio, la Regione potrebbe essere d'aiuto in questo senso. Sono tante le misure che si potrebbero mettere in campo, come per esempio il *bonus retrofit* per la conversione del motore termico in un motore elettrico;

termovalorizzatori, in tutta l'Italia ce ne sono 31, di cui 26 sono nel Nord d'Italia, nella Pianura padana. Visto che stiamo già abbastanza bene, i termovalorizzatori li mettiamo tutti lì: nella Regione Lombardia ce ne sono 13. Occorrerebbe una politica di graduale dismissione, anche abbastanza rapida, e riconversioni di questi impianti, anche perché è evidente che noi stiamo bruciando i rifiuti di qualcun altro, perché non è possibile che bruciamo i nostri.

in realtà le azioni che questo Governo avrebbe potuto mettere in campo a livello di principi guida per le Regioni verso la soluzione del problema non ci sono state; abbiamo addirittura inserito il punto strategico dell'aeroporto di Malpensa. Una volta tanto che si era riusciti a preservare il suolo, che assorbe anidride carbonica, salvando la brughiera, adesso trasformiamo l'aeroporto di Malpensa in un punto strategico e ho come l'impressione che quella brughiera stia correndo seri rischi. Sappiamo che la direttiva europea sulla qualità dell'aria approvata il mese scorso dal Parlamento europeo si propone di avvicinare i limiti di concentrazione dei principali inquinanti a quelli previsti dall'Organizzazione mondiale della sanità, probabilmente la procedura di infrazione non si arresterà, perché questi limiti cambieranno. Tuttavia le Regioni del Nord, quelle più coinvolte, si sono opposte all'approvazione di questa

di fronte alla tutela della salute non c'è portafoglio che tenga. È quindi evidente che la visione di questa maggioranza rispetto alla tutela della salute e dell'ambiente mi lascia alquanto perplessa: non si può anteporre l'interesse economico alla tutela della salute dei cittadini.

che si proponeva di riportare al pubblico la funzione di programmazione e di pieno controllo dell'erogazione dei servizi sanitari. Il problema ulteriore è che le persone nel Nord Italia si ammalano a causa della presenza di inquinamento; tuttavia, per accedere al servizio sanitario - come ben sapete - la Regione Lombardia ha delle forti criticità: mancanza di infermieri, problemi di pronto soccorso, sanità principalmente privata. Il costo della vita nelle Regioni del Nord è altissimo e un lavoratore medio non può permettersi la sanità privata, pertanto rimane condannato ad aspettare anni per essere curato da quella malattia che gli è stata causata dalla presenza dell'inquinamento atmosferico. In conclusione, quello che mi lascia perplessa è l'ordine delle priorità di questo Governo, il fatto che non condivida appieno il processo verso la transizione ecologica, ma sarà costretto a farlo e purtroppo, quando capirà come dovrà comportarsi sarà troppo tardi.

a volte abbiamo raggiunto nel corso dell'esame della conversione in legge di questo decreto hanno effettivamente rasentato quelli tipici della battaglia politica e forse forse in alcuni momenti sarà parso all'esterno ai non addetti ai lavori che ci fosse un confronto fra oscurantisti, ovvero quei conservatori che non vogliono assolutamente che si cambi nulla, che avvenga avvenga il naturale processo di modernizzazione del Paese, e gli speculatori, quei classici investitori che non sono invece sensibili ai problemi ambientali e alla salute delle persone. vorrei riportare nell'alveo della normalità e del confronto dialettico e democratico la trattazione di un importante argomento qual è quello di misure che vanno nel senso, invece, di apprezzare quale possa essere la migliore qualità dell'aria, il miglior stile di vita, perché oggi la cura della persona, l'attenzione verso l'alimentazione, verso gli ambienti nei quali si vive è certamente fra i primi problemi a cui la comunità, e quindi anche la politica, è tenuta a fare molta attenzione.

con questo provvedimento si va a dare una risposta, ahimè, ai ritardi con i quali il Paese ha affrontato delle richieste che ormai provengono da un ambito comunitario al quale abbiamo deciso di partecipare. Siamo pienamente coscienti degli impegni che incombono:

acuite da particolari fattori come quello orografico e come quello eolico, dove ci sono delle situazioni che, ahimè, alimentano la permanenza e non facilitano la dispersione del cosiddetto particolato, che in parte è dovuto a eventi e fenomeni naturali e in parte viene immesso

Ebbene, si accusano la politica, il Governo attuale di non fare o si accusano le Regioni che magari sono in ritardo, ma io vorrei citare il fatto che lo scopo di questo provvedimento è proprio quello di valorizzare un percorso iniziato da quell'accordo di programma tra il tra il Ministero dell'ambiente e le Regioni interessate che nel 2017 ha messo in corsa queste Regioni per andare verso un sistema di valutazione omogenea della qualità dell'aria e dell'ambiente sulla base di metodi che possano consentire una risposta omogenea e naturalmente ha impresso un'azione per disciplinare e mantenere la qualità dell'aria e dell'ambiente laddove questa è buona e migliorarla negli altri casi.

drammatici, come il periodo estivo, oppure nei momenti in cui fa comodo a qualcuno, specie i criminali del settore, che purtroppo proliferano proprio grazie a queste politiche del «no» sull'impiantistica. Ebbene, vorrei sottolineare come auspichiamo lo sviluppo di una linea politica ecologica che sia ispirata da criteri liberali, rigorosamente laica, che assuma come base per le sue scelte la necessità di garantire uno sviluppo scientifico che consenta una rapida diffusione delle tecnologie più accreditate e verificate, naturalmente senza vincoli di utilizzo derivanti da obblighi normativi, ma consentendo ai criteri di mercato e all'accessibilità economica di far sì che queste tecnologie vengano poi poi definite le migliori. È evidente che la questione della mobilità nelle nostre città non si risolve con il solo cambio a favore dell'auto elettrica, ma attraverso una pianificazione di nuove infrastrutture per dare alle città una mobilità pubblica sostenibile. È il motivo per cui iniziamo ad applicare certe normative partendo dai centri urbani maggiormente dimensionati, che possono garantire ai cittadini una circolazione alternativa pubblica adeguata a non interrompere la mobilità delle persone e soprattutto delle merci, visto che questo provvedimento riguarda anche i veicoli destinati al trasporto delle merci. Altrimenti, dovremo scontare un indecoroso fenomeno del «no» a ben sperimentate tecnologie, come quella per lo smaltimento dei rifiuti, e sono queste impostazioni pericolose che noi respingiamo. Le vorrei definire un po' da cultura da «Fahrenheit 451», quel famoso romanzo da cui poi fu tratto uno splendido film, nel quale, in un'epoca in cui i *mass media* danno una disponibilità apparente, concedendo ampio spazio all'accesso alle fonti culturali, gli stessi tendono poi ad oscurarne l'importanza, convogliando l'attenzione di massa su orizzonti del tutto diversi. Vorrei dire che noi certamente non bruciamo i libri,

Risalgono a sette-otto anni fa: era nel 2015. Il primo è Bruno, un ingegnere che lavora in una grande società italiana di impiantistica. Lavora in tutto il mondo, erede di quella grande tradizione del saper fare italiano, e quando nel 2015 una grande multinazionale cinese, che sta lavorando - come sappiamo - all'infrastrutturazione del Continente africano, lo chiama per fargli una proposta di lavoro,

lorda che è più che doppia rispetto a quella che guadagna in Italia. Gli offrono una casa per sé e per la sua famiglia, offrono a sua figlia che ha vent'anni non soltanto il pagamento delle più prestigiose università di Pechino, ma anche l'alloggio e tutte le coperture sanitarie e sociali. Dopo che discute con la sua famiglia e decide di accettare questa proposta, si reca a Pechino; torna dopo quattro-cinque giorni e dice alla sua famiglia di aver rifiutato questa offerta e che aveva già deciso. L'altra storia è quella di Giorgio, anche lui ingegnere genovese. Lavorava già all'epoca in un grande centro di ricerca europeo, ricercatore stimato con un *H-index* molto elevato, con pubblicazioni internazionali; anche lui viene chiamato da un centro di ricerca di Pechino, gli offrono una RAL molto superiore a quella che riceveva in Europa, gli offrono casa, gli offrono la copertura sanitaria e la copertura scolastica per i due figli piccoli. Anche lui decide di andare perché è un'offerta economicamente molto vantaggiosa; anche lui, dopo essere stato a Pechino, torna indietro dopo pochi giorni e annuncia di aver rifiutato. Qual è l'elemento comune di queste due storie? Entrambi sono stati a Pechino e hanno visto la nube di smog che c'era nella regione dell'Hebei; entrambi hanno deciso che non c'era non c'era prezzo per portare loro e le loro famiglie a vivere in quel contesto inquinato e potenzialmente pericoloso per la loro salute e quella delle loro famiglie. Voglio ribadirlo perché troppo spesso ho sentito in questa discussione parlare di ambiente e di sviluppo economico come se fossero in contrapposizione. Ma la storia moderna è diversa: noi ricerchiamo un nuovo modello di sviluppo perché solo con un nuovo modello di sviluppo compatibile con la qualità della vita, con la qualità dell'aria e con la qualità dell'ambiente possiamo avere un futuro, dal punto di vista economico, per il nostro Paese. credo che ben venga se un Governo, di fronte alla possibilità di un'infrazione per lo sforamento dei limiti di inquinamento, decide di adottare misure urgenti

i problemi derivanti da questi inquinanti; non si forniscono tempistiche che sollecitano provvedimenti urgenti; come hanno ricordato i colleghi, si impedisce alle Regioni di avviare provvedimenti urgenti, dilazionando in avanti la data dalla quale si può partire per fare provvedimenti urgenti; urgenti; non si condividono nemmeno gli obiettivi con le stesse Regioni interessate. Stiamo votando un decreto con il parere negativo della Conferenza Stato-Regioni che - lo ricordo alla maggioranza - in questo momento è a maggioranza centrodestra. quindi un provvedimento che viene vissuto semplicemente come un atto dovuto, che però non aiuta a superare il problema; al contrario, vuole sostenere, per ragioni elettorali, alcune Regioni inadempienti a non agire, superando le richieste europee con espedienti burocratici. Servirebbe ben altro: servirebbero scelte strategiche di politica industriale e risorse strutturali per il trasporto pubblico locale e per la mobilità pubblica. Abbiamo provato Abbiamo provato a presentare emendamenti sul trasporto pubblico locale e per rafforzare il *bonus* trasporti, ma nessuna risposta è stata data dal Governo. Servirebbe una cura del ferro e un nuovo piano di politica industriale che guardi a quello di cui realmente il Paese ha bisogno. Invece state semplicemente rimandando il problema. Pensate che questa furbizia di andare più in avanti e di rispondere all'Unione europea con una non risposta possa risolvere il problema, ma quando si mette la sabbia sotto il tappeto non si risolvono i problemi. Dobbiamo restituire al Paese un ambiente più sano, moderno, capace di salvaguardare la salute dei cittadini, capace di essere competitivo nell'attrarre e conservare le competenze. È chiaro ormai che di questo non volete occuparvi. All'Italia serve una politica industriale che ci permetta di competere con le grandi economie occidentali, che punti su tecnologie digitali, sulla transizione ecologica, sulla centralità del benessere dei cittadini. Credo che con il decreto-legge in esame, con le vostre politiche e con l'annunciata legge di bilancio voi non stiate affrontando questo problema. Questo è il tema da mettere al centro dell'agenda; non lo state facendo e per questo noi voteremo convintamente no a questo decreto. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il decreto-legge in discussione quest'oggi in Senato dimostra la volontà del Governo di tutelare la salute pubblica contrastando l'inquinamento atmosferico. Sebbene i dati sulla qualità dell'aria della nostra Nazione ci dicono che negli ultimi dieci anni si registra un miglioramento dei valori, in alcune parti del territorio nazionale permangono forti criticità.

coesistono condizioni meteoclimatiche e orografiche, che in particolari mesi dell'anno, favoriscono l'accumulo di elementi inquinanti nell'atmosfera. Su quest'area, che comprende le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, il legislatore è già intervenuto in passato con la legge 88 del 2009, prevedendo l'adozione di specifiche strategie di intervento, anche attraverso un maggior coordinamento tra le Regioni interessate. In attuazione di questa legge sono stati firmati anche diversi accordi di programma: in particolare ricordo quello del 2017, finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano, che prevedeva per le Regioni interessate una serie di interventi comuni da porre in essere nei settori particolarmente inquinanti, oltre a quelli previsti nei piani della qualità dell'aria. altresì che per queste Regioni sono stati attivati anche programmi di finanziamento per promuovere il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale. esame interviene nuovamente sul problema atmosferico del bacino padano e ha anche il compito di assicurare l'esecuzione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea. Nei confronti dell'Italia, infatti, sono pendenti tre procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea per la cattiva applicazione della direttiva sulla qualità dell'aria. Nello specifico, è stato contestato che nel periodo dal 2008 al 2017 in alcune parti del territorio italiano si è registrato in maniera sistemica e continua il superamento dei valori limite di inquinamento. Con il decreto-legge in esame quindi le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono obbligate a provvedere entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore all'aggiornamento dei rispettivi piani della qualità dell'aria. Inoltre, in attesa dell'aggiornamento dell'aggiornamento dei piani della qualità dell'aria, viene concessa alle Regioni la possibilità di limitare, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo, la circolazione stradale per le autovetture e i veicoli commerciali categorie N1, N2 e N3, alimentati con diesel, di categoria euro 5, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.

infatti data la centralità al ruolo delle Regioni proprio con l'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria, quale strumento principe per intervenire con determinazione sull'inquinamento atmosferico. piani prevedono fasi ben precise di programmazione degli interventi, di valutazione dei dati delle emissioni e delle condizioni climatiche, di applicazione degli interventi e di verifica dei risultati raggiunti. Sbaglia chi sottovaluta questo aspetto, come sbaglia chi sottovaluta le tante azioni che questo Governo sta portando avanti sul tema della qualità dell'aria. Ieri, durante la discussione generale, il collega Rosa ha ricordato l'incremento di 30 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 del Fondo per le misure relative ai trasporti, alla mobilità sostenibile, alla combustione domestica della biomassa e all'efficientamento energetico. Dobbiamo ugualmente ricordare le azioni messe in campo dal ministro Lollobrigida per incentivare l'agricoltura sostenibile. Il Governo sta mostrando una grande attenzione alle tematiche ambientali, ma c'è un altro modo

gratuitamente, a un costo sociale e ambientale che vi portate sulla coscienza. di stabilire come orizzonte temporale la data del 1° ottobre 2024 per eventuali limitazioni alla circolazione è stata oggetto di confronto in Commissione; una scelta che il Governo ha ampiamente motivato all'interno della relazione, dove viene specificato testualmente che tale scadenza tiene conto delle criticità legate alla indisponibilità dei materiali necessari alla produzione di batterie di veicoli elettrici in grado di assicurare una tempestiva sostituzione dei veicoli Euro 5. pone in evidenza, a motivazione della decisione, un tema che non è affatto scontato, e cioè quello della sostenibilità delle scelte, ossia la capacità di una norma di produrre effetti concreti sui territori, valutando le ricadute che questi possono comportare nel tessuto economico e sociale. Il tema della sostenibilità della scelta è di grande attualità e riguarda non solo il bacino padano ma anche molte altre realtà. Si inserisce in questo contesto - e non è affatto fuori tema - l'accorato appello che la senatrice Mennuni ha voluto

la scelta della Giunta Gualtieri sulla gigantesca area ZTL che dovrebbe entrare in vigore dal 1° novembre, che mette in difficoltà l'intera città, i lavoratori e i cittadini (circa 800.000 persone) che non hanno a disposizione un'auto di ultima generazione. Su questo tema non si può evidentemente far finta di nulla. Bisogna necessariamente aprire una riflessione e mostrare una sensibilità diversa. Più volte ho sentito esponenti dell'opposizione dichiararsi, anche durante il dibattito, favorevoli al principio che la transizione energetica non debba essere ideologica; un principio assolutamente fondamentale, un principio giusto, che però ha bisogno di essere sostenuto, non solo con le parole, ma anche con i fatti. Francamente sono rimasto sono rimasto perplesso nel leggere alcuni emendamenti portati all'attenzione della Commissione dall'opposizione, perché confliggono con la dichiarata volontà di non ideologizzare il tema della transizione. In Commissione è stato, ad esempio, proposto dal MoVimento 5 Stelle di estendere la possibilità di limitare la circolazione stradale a tutte le autovetture e ai veicoli commerciali alimentati con motori endotermici, non ritenendo evidentemente sufficienti le limitazioni alle auto Euro 5: mi sembra proprio che le preoccupazioni del mondo economico, dei cittadini e di molte istituzioni sulla transizione non interessino alle opposizioni. Invito i senatori del centrosinistra a riflettere su quanto è accaduto anche al Parlamento per quanto riguarda l'approvazione degli *standard* delle auto Euro 7, dove le sinistre e i verdi, che avevano dimostrato un approccio ideologico sulla materia, sono stati sconfitti da posizioni più pragmatiche, che hanno dato vita a un'ampia maggioranza, che ha portato a concedere ai produttori di auto e furgoni un periodo di tolleranza temporale più ampio prima di conformarsi ai nuovi *standard* di emissioni. La stessa identica cosa è successa qualche giorno fa per quanto riguarda le case *green*. Voglio essere chiaro: la transizione energetica è una priorità del Governo Meloni. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di tutelare la salute pubblica dall'inquinamento atmosferico. Siamo convinti della necessità di incentivare il trasporto delle merci su ferro, in alternativa a quello su gomma. Crediamo in uno sviluppo sostenibile, che sia in grado di trovare un nuovo equilibrio tra natura e uomo; una sostenibilità che, però, deve essere autenticamente sostenibile (e il gioco di parole è voluto), perché se così non fosse sarebbe destinata a rimanere un mero esercizio di retorica, condannato a non produrre alcun effetto.

che il decreto-legge vada proprio in questa direzione ed è per questo che, a nome di Fratelli d'Italia, annuncio il voto favorevole

è volto a segnalare un fatto di una gravità inaudita, che comprime i diritti dei consiglieri comunali e di conseguenza dei cittadini e che ha trasformato il Comune di Vittoria in un *bunker* e non in una casa di vetro, come pure prevede la norma sulla trasparenza degli enti locali. Infatti il Comune di Vittoria, retto da una Giunta del PD e dal sindaco Francesco Aiello, ha negato un'istanza di accesso agli atti depositata lo scorso 28 settembre 2023 dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Valeria Zorzi. La consigliera aveva chiesto la copia della relazione finale depositata dagli ispettori regionali sull'attività amministrativa del Comune di Vittoria. Infatti il Comune di Vittoria, Presidente, per irregolarità gestionali e amministrative, più volte denunciate anche dai consiglieri di Fratelli d'Italia, ha subito diverse ispezioni regionali disposte dall'Assessorato regionale agli enti locali, che ha profilato, nero su bianco, delle attività illegittime e reiterate. L'ente comunale, in data 6 ottobre 2023, ha negato l'accesso agli atti e quindi non ha consegnato la relazione degli ispettori, con la seguente motivazione: la relazione è oggetto di esposto in procura. Diniego avallato persino da una relazione del capo di gabinetto del sindaco. Il predetto diniego costituisce una gravissima violazione del diritto del consigliere comunale all'accesso agli atti, espressamente disciplinato dall'articolo 43, comma 2, del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000,

«Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»